a chi ha la responsabilità della sua applicazione con riferimento al maxiemendamento presentato dal Governo. Non intendo assolutamente riprendere le questioni svolte ieri, ma voglio ribadire, di fronte

circostanza aveva tra l'altro indotto il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, all'epoca dell'approvazione della riforma dell'ordinamento giudiziario, a richiamare le Camere

costituivano il cuore della delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Oggi abbiamo un disegno di legge che si compone di 1.365 commi.

per cui, se volessimo contare i commi che compongono il maxiemendamento, sono convinto che supereremmo, forse, quota 2.000. È vero, signor Presidente, che nel passato

1.365 commi, che rendono il testo difficilmente conoscibile all'origine già per

le fiducie richieste alla Camera - ed una di queste riguarda la finanziaria - sono pari, o quasi, a quelle richieste al Senato. Anche sulla fiducia c'è una degenerazione. È inutile che i colleghi richiamino le 40 fiducie del Governo Berlusconi in cinque anni. Se si dovesse applicare la media di queste fiducie, supereremmo, nei cinque anni di legislatura, magari con più Governi (ed io lo auspico), le 100 e più fiducie. Credo che questa china non possa esser

a tutela non solo della Costituzione e del Regolamento, ma anche di chi deve applicarlo. In mancanza di norme certe mi rendo conto che chi deve applicare il Regolamento si trova sottoposto a spinte e controspinte che possono incidere sulla sua decisione

ad una deliberazione della Giunta che è datata e risale a diversi lustri fa. Quando fu adottata quella deliberazione, il contesto era molto diverso e nessuno avrebbe mai immaginato che si sarebbe arrivati ad un maxiemendamento come quello oggi in votazione.

nella notte siano state modificate alcune tabelle. Ad esempio, ieri avevo denunciato come sul Fondo di finanziamento ordinario dell'università fossero appostati appena 13 milioni di euro.

della consegna e della distribuzione del maxiemendamento, che era stato già comodamente pubblicato sul sito del «Corriere della Sera» un'ora prima che noi senatoriricevessimo il testo.

Credo che se ciò accadesse all'interno del Senato, se cioè un funzionario, in ragione del suo servizio, distribuisse qualcosa fino allora coperto da segreto, verrebbe giustamente appeso al pennone (e credo potrebbero farlo anche altrove). Inoltre, trovo disdicevole che venga consegnato un testo a fianco il commento e lo *sponsor* dell'emendamento. Posso accettare che il Governo presenti un testo, ma che la cosa sia consigliata dal dottor Massicci francamente mi disturba. Così come mi disturba leggere che un emendamento, che è stato inserito, sia ancora da rivedere, perché non capisco se quello è definitivo oppure se devo immaginare una modifica successiva da parte

politica e civile. Essa - a mio avviso - segna un decadimento dei rapporti non solo istituzionali, ma anche civili. Ci sono molti mondi che stanno

- nessuno si scandalizzi - che le vacanze interessano tutti. Se andate a guardare le leggi del vecchio Giolitti, noterete che sono tutte targate alla vigilia delle vacanze di Natale oppure il 2 o il 3 agosto.

per serietà; altrimenti personalmente, forse data anche la mia età, non sono in condizioni di capire bene quello su cui voteremo.

l'articolo di una legge costituzionale con una legge ordinaria. Ma poi ci è stato fornito l'articolo 63 dello Statuto

sia pure per legge costituzionale, si possa stabilire che quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 116 possa essere superato. Ho dato

Presidente, non ripeterò le argomentazioni già svolte dagli illustri colleghi che mi hanno preceduto.

annunciato all'Assemblea, chiedo al presidente Morando di informare l'Assemblea stessa sul dibattito che si è svolto presso la Commissione bilancio, dopo le indicazioni che sono emerse, in maniera alla fine pressoché unanime, nella discussione in Aula di ieri pomeriggio.

esame che ci è stato sollecitato per i profili di copertura del complesso delle norme e di ciascuna delle norme in esso contenute, oltre che per il rispetto del cosiddetto contenuto proprio della legge finanziaria, così come fissato dalla legge di contabilità, questa volta è stato reso, signor Presidente, più agevole dalla scelta - lo dico a futura memoria memoria - proposta dalla Commissione e accettata dal Governo e dal relatore di presentare tutti gli emendamenti, compresi quelli del Governo e del relatore, al momento del termine della discussione generale in Commissione e nei limiti temporali imposti all'attività emendativa dei senatori. Ciò ha reso possibile un esame più attento delle relazioni tecniche relative alle relative alle proposte del Governo e del relatore, aggiornate via via in sede di presentazione di eventuali riformulazioni degli emendamenti stessi. Tanto che, signor Presidente, nelle ore scorse è stato possibile vagliare le norme contenute nel testo dell'emendamento 1.1000 alla luce delle vecchie relazioni tecniche, confrontandole e integrandole con quella nuova allegata all'emendamento 1.1000. Ne emerge, signor Presidente, allo stato degli atti, un giudizio di corretta copertura della legge finanziaria, così come riscritta attraverso l'emendamento 1.1000. Segnalo ai colleghi senatori e a lei, signor Presidente, che vi è una serie di commi aggiuntivi, accoglitivi di emendamenti parlamentari, per i quali è prevista copertura sulle tabelle che che sono appositamente rideterminate (in particolare la tabella C, ma anche la tabella A). Si tratta dei commi 640 e 605, corrispondenti a parti dell'emendamento 18.1550; del comma 579, corrispondente al comma 259-*bis* dell'emendamento 18.600; del comma 642, in parte corrispondente all'emendamento della senatrice Levi-Montalcini;

questi commi perché la verifica della loro corretta copertura non è immediata, come per gli altri, ma dev'essere compiuta con riferimento alla rideterminazione delle tabelle. Per quel che vale, questa verifica, compiuta prima dal sottoscritto in collaborazione con gli uffici e poi dalla Commissione, effettuata - ripeto - con una collaborazione tecnica adeguata, conduce a concludere che anche tali commi sono correttamente coperti. Il prospetto di copertura, comprensivo degli effetti dell'emendamento 1.1000, rimodula sia gli oneri da coprire, sia i mezzi di copertura, determinando nel complesso un minore utilizzo del miglioramento del risparmio pubblico, rispetto a quanto avveniva ad opera del testo approvato dalla Camera. Esso indica i seguenti oneri da coprire: 24.245 milioni per il 2007; 26.481 milioni per il 2008; 26.494 milioni per il 2009. Gli effetti dell'emendamento 1.1000 sono indicati, colleghi, in 750 milioni per il 2007; 729 milioni per il 2008 e 549 milioni per il 2009 di maggiori spese nette (quelle recate cioè dalle scelte di spesa modificative delle scelte di spesa che ci vengono dalla Camera), a fronte di 901 milioni, 591 milioni e 583 milioni di maggiori entrate nette. Vengono inoltre ridotte le spese di cui alle tabelle A e C e vengono aumentati i decrementi di cui alla tabella E sul lato delle entrate. Il margine complessivo, cioè il frutto complessivo dell'emendamento così come presentato, aumenta dunque da 18.045 milioni a 18.416 milioni, nell'anno 2007, con un miglioramento di 371 milioni; da 27.728 a 27.844 milioni, nel 2008, con un miglioramento di 116 milioni; e da 42.613 milioni a 43.077 milioni, nel 2009, con un miglioramento di 463 milioni. I mezzi di copertura, indicati nel prospetto in esame, risultano pertanto adeguati per ciascuno degli anni del triennio. In particolare si segnala che, nel secondo anno del triennio, l'effetto netto dell'emendamento 1.1000, in termini di aumento degli oneri correnti da coprire, supera le maggiori entrate determinate dallo stesso emendamento, ma i mezzi di copertura necessari derivano dai tagli effettuati sulle tabelle A e C. su questo punto, che riguarda il prospetto di copertura nel suo complesso, i colleghi dell'opposizione, durante la discussione che si è svolta in Commissione,

La prima osservazione riguarda quella che chiamerei la credibilità e la realizzabilità delle maggiori entrate recate a copertura di spese certe. certe. I colleghi dell'opposizione sostengono che la parte delle maggiori entrate che deriva da interventi per l'istituzione di nuovi giochi o per la modifica della regolazione dei giochi,

a fronte invece di spese certe. Ritengono quindi che su questo punto il prospetto di copertura sia tecnicamente redatto in maniera perfetta, ma che in realtà «nasconda» maggiori entrate non realizzabili, e che saranno non realizzate, così determinando di fatto, almeno per questa parte, un certo livello di scopertura

a proposito di alcune norme dello stesso, e relativa all'utilizzo, a fini di copertura di maggiori spese correnti (non particolarmente rilevanti, ma in ogni caso presenti nel testo), nel testo), delle minori spese correnti derivanti da riduzione della spesa per interessi, in forza di interventi di riduzione dello *stock* del debito pubblico che si realizzino attraverso un complesso di operazioni, tra cui si segnala, in particolare, quella relativa ai cosiddetti conti

di quella discussione - segnalano che tecnicamente, e anche politicamente, a loro giudizio, c'è un'incertezza di valutazione sulla correttezza dell'uso di queste risorse per coprire oneri correnti. La terza osservazione dei senatori dell'opposizione su questo punto, sul prospetto di copertura in generale, è quella relativa, sempre a loro giudizio, ad una non perfetta o non compiuta valutazione da parte del Governo

la copertura degli oneri attraverso tagli orizzontali della tabella C è certamente corretta dal punto di vista tecnico, quindi *nulla quaestio* sul prospetto di copertura in quanto tale,

sulla base dell'emendamento 1.1000. Alcune valutazioni necessariamente si incroceranno con problemi di copertura.

In particolare, le segnalo in primo luogo (perché su questo punto c'è un'assoluta unanimità della Commissione) il comma 923 dell'emendamento al nostro esame, il quale proroga i termini per l'esercizio della delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose. Mi riferisco alla legge n. 32 del 2005, una legge di delega. Il comma 923, signor Presidente, è identico al capoverso 502-*septies* dell'emendamento 18.144 del Governo, io ho dichiarato inammissibile in sede di discussione in Commissione perché proroga i termini per l'esercizio di una delega. È fuori discussione, a mio giudizio, che questo emendamento fosse effettivamente inammissibile (difendo quindi la correttezza della mia scelta per il dibattito in Commissione), perché, se è vietato iscrivere

nella legge finanziaria anche soltanto con una proroga dei termini per l'esercizio della delega: infatti, per omogeneità di trattamento, si tratterebbe di una norma di delega, sia pure attraverso il mero allungamento dei termini. segnalo questo per eventuali sue determinazioni. Il parere della Commissione è unanime sul fatto che sarebbe meglio che tale norma venisse espunta dal testo. I senatori Vegas e Ripamonti hanno segnalato che i commi 922 e 945 conservano in bilancio somme perenti. Ciò, signor Presidente (lo dico come cosa pacifica e convenuta da tutta la Commissione), costituisce una violazione della norma di contabilità e, di fatto, implicitamente ne contiene una modifica. Voi sapete, colleghi senatori, che modifiche della legge di contabilità non sono ospitabili all'interno della legge finanziaria. Tuttavia, signor Presidente, mentre le faccio questa segnalazione, le debbo anche dire che in proposito, forse per mio errore (e se lei in tal senso valuterà, naturalmente non me la prenderò a male), mi a male), mi sono regolato circa l'ammissibilità di queste due norme, già contenute negli emendamenti presentati in Commissione: essendomi proposto il tema della loro ammissibilità per le ragioni che ho già esposto, mi sono regolato nel senso di valutare che norme di questo tipo, di fatto modificative della legge di contabilità, erano contenute nel testo che ci giungeva dalla Camera, essendo state là evidentemente considerate ammissibili. Mi sono posto di conseguenza - lo dico sinceramente - un problema piuttosto complicato da risolvere: potevo io alla Commissione bilancio del Senato disporre l'inammissibilità di un testo assolutamente identico, sotto il profilo formale (quello di cui mi stavo occupando, cioè il rispetto del divieto di introdurre modifiche alla legge di contabilità nella finanziaria), ad ad un testo di legge che ci giungeva dalla Camera con modifiche al suo interno assolutamente identiche nella forma e nella sostanza alla norma che mi stavo apprestando a dichiarare inammissibile? Pensa che ti ripensa, alla fine, li ho dichiarati ammissibili. Il Governo non ha, quindi, nessuna responsabilità se, avendo preso atto della loro ammissibilità, ha inserito quelle norme nel testo dell'emendamento 1.1000. Segnalo questa situazione ed anche che il mio parere resta quello che mi ha ispirato nello scegliere a favore dell'ammissibilità. Presidente, sarò pronto a considerare assolutamente fondata tecnicamente una sua eventuale scelta di tipo diverso, nel senso che posso aver sbagliato io e potrebbe fare correttamente o più correttamente lei, dichiarando quelle norme inammissibili. Le ho segnalato le due norme del caso e tanto dovevo, anche se non le sfuggirà che, in caso di dichiarazione di inammissibilità, un qualche problema nei confronti dell'altro ramo del Parlamento obiettivamente insorgerebbe, perché ci staremmo regolando in modo diverso. Tuttavia, sostengo

state quelle presenze nel testo della Camera non avrei avuto dubbi nel dichiarare inammissibili questi due commi - lo dico subito - già in sede di discussione in Commissione. inoltre, signor Presidente, due problemi che non hanno direttamente a che fare con la copertura, ma forse un po' con il contenuto proprio: si

giacché interviene su un soggetto privato i cui organi sono espressione di diversi soggetti istituzionali. Alla Commissione bilancio è apparsa assolutamente consigliabile una decisione di espunzione di questa norma dal testo, ma naturalmente stiamo dando un consiglio, non stiamo disponendo alcunché. La ragione di questa espunzione, ripeto, sta nel difficile rapporto tra la norma così com'è e il carattere dell'organismo su cui si sta intervenendo. Le ricordo,

di considerare ammissibili interventi su organi di enti ed istituzioni che fossero di diretta emanazione e di esclusiva competenza dello Stato centrale e non anche di organismi come quelli al nostro esame, che sono il frutto del concorso di diverse istituzioni. Pertanto, intervenire d'autorità con la legge su un'istituzione sostanzialmente privata, per modificare il consiglio di amministrazione di un organismo che è espressione di soggetti istituzionali assolutamente diversi, ci

e quindi inaccettabile. Abbiamo discusso lungamente sul testo e abbiamo alla fine

da quell'emendamento la copertura (che non è necessaria, perché la relazione tecnica ha già modificato le tabelle, prevedendo la copertura della norma riferita alla sola Provincia di Bolzano), a quel punto tra relazione tecnica e testo ci sarebbe coerenza e non si porrebbero problemi

formale legittimità, che è stata documentata dal Governo attraverso il riferimento ad una legge. Comunque, su questo non sono in grado di riferire una discussione in Commissione che non c'è stata; segnalo, semplicemente, la presenza di questa

legittimamente, ma a mio avviso impropriamente, a considerare con un eccesso di rigidità l'esigenza che abbiamo riscontrato, punto per punto, che tutte le norme inserite nell'emendamento 1.1000, senza eccezione, cioè tutte le norme modificative del testo ricevuto dalla Camera, trovassero fondamento per materia in emendamenti presentati in Commissione. Nel corso della discussione non abbiamo potuto trovare una sola norma che non abbia questa caratteristica: se c'è una disposizione modificativa del testo che ci proviene dalla Camera presentata nel testo dell'emendamento 1.1000, quella norma ha un fondamento per materia in un emendamento presentato in Commissione, senza alcuna eccezione. Naturalmente, invece, non è detto che la norma contenuta nell'emendamento 1.1000, corrispondente per materia all'emendamento parlamentare presentato in Commissione, lo sia in modo talmente perfetto da coincidere in ogni suo aspetto. aspetto. Peraltro, un'interpretazione di questo tipo sarebbe del tutto ultronea, perché nei lavori della Commissione sistematicamente si parte da un emendamento e si provvede poi ad eventuali riformulazioni da parte del relatore o del Governo. Quindi, è ovvio che la nostra verifica, per come io l'ho interpretata, doveva riguardare la presenza di emendamenti su quella materia, non la presenza di emendamenti identici, a pena di nullità, dei testi di norma presentati dal Governo nel suo emendamento 1.1000. Da questo punto di vista,

Ci sono, invece, molte norme che, trovando questo fondamento, hanno poi subito una riformulazione, ma a me sembra che ciò sia perfettamente corretto. *(Applausi

valutato il suo lavoro e il merito di quegli emendamenti, propone che il Governo sia autorizzato a integrare il testo con queste due norme che - ripeto - sono

che la Commissione unanimemente riconosce non essere state inserite nel testo dell'emendamento 1.1000 soltanto per un mero errore materiale compiuto in questo caso dal Governo (qualche errore l'ha compiuto anche il Governo), diversamente da quelli precedenti che invece sono errori miei.

sottoposto all'attenzione dell'Assemblea nel mio intervento precedente. Devo anche aggiungere che nelle tabelle fornite dal Servizio Studi del Senato risulta, sempre con riferimento all'università, un taglio di risorse

su quali siano i dati reali, perché siano cambiati rispetto al testo originario e quando siano cambiati rispetto ai testi distribuiti alla Commissione e alla Presidenza del Senato;

l'intervento degli organi costituzionali nel processo legislativo. Sono emerse alcune valutazioni di carattere costituzionale estremamente delicate che la Commissione affari costituzionali non ha potuto o forse voluto (naturalmente non è nella mia disponibilità verificarlo) approfondire. Le modifiche, indubbiamente particolarissime, degli Statuti non solo della Sardegna, ma anche del Friuli-Venezia Friuli-Venezia Giulia (commi 836 e 949) indubbiamente hanno un riferimento a norme degli Statuti regionali, ma non possono essere liquidate

quale sarebbe estremamente originale se mantenessimo o ritenessimo ancora in vigore norme di Statuti speciali che consentono a leggi ordinarie, sentita la Regione (tra l'altro, un soggetto così anonimo), di modificare alcune parti di Statuti; poi abbiamo norme costituzionali che si applicano a tutte le Regioni dove c'è un procedimento ben preciso di approvazione e di modifica degli Statuti. Tale questione non può essere risolta in maniera così sbrigativa. Mi rendo conto dei problemi di questa sessione,

che hanno lo stesso grado delle leggi ordinarie, com'è una legge finanziaria e una qualsiasi legge approvata dalla Camera e dal Senato, ma che contengono in sé delle norme dettate verso il legislatore, ossia verso i soggetti che devono presiedere al rispetto delle regole nella produzione delle norme legislative. Questo vale per la legge di contabilità, ma vale anche per lo Statuto del contribuente. Se vogliamo che si rispetti quella volontà, occorre che chi è chiamato a far rispettare le regole procedurali faccia presente, in ogni momento, che vi sono leggi di grado superiore, se non formalmente

di leggi che devono considerarsi di rilevanza assolutamente costituzionale. Signor Presidente, abbiamo lavorato tutta la notte per dare la consulenza che lei ha chiesto alla Commissione bilancio sul testo che è stato distribuito ieri alle ore 19,15;

nella versione che ci è stata consegnata ieri alle ore 19,15, risulterebbero diverse dalle tabelle del Servizio Studi del Senato distribuite questa mattina. È opportuno che il Governo chiarisca questa differenza che non poteva emergere in Commissione, perché ci riferivamo al testo che ci era stato formalmente consegnato ieri sera.

di interesse particolare. La questione che volevo porre è quella relativa all'ultima segnalazione fatta dal presidente Morando, consentire consentire cioè al Governo di inserire due emendamenti, quello relativo ai *broker* assicurativi e quello riferito alle Olimpiadi di Torino

se si acconsentisse a questa variazione in corso d'opera, per cui pretenderei, in questo caso, di vedere quale delega ha il ministro Chiti per poter fare ciò. credo che quanto riferito dal presidente Morando sia molto corretto. Ha fatto un'analisi puntuale di quanto è avvenuto in Commissione bilancio,

che possa essere modificato, perché la Commissione è d'accordo sulle due norme richiamate anche dal senatore Paravia, andiamo verso uno stravolgimento del procedimento legislativo.

Il comma 1365 - non mi stancherò di richiamarlo - afferma: «La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2007» - questo è corretto perché la legge finanziaria è la legge che riguarda l'esercizio dell'anno successivo «ad eccezione dei commi 538-*bis*, 538-*ter*, 538-*quater*, 538-*quinquies*, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge». Queste norme sono riferite chiaramente al bilancio delle Ferrovie dello Stato e sono un trucco contabile che viene operato con questa finanziaria, che si collega anche alla vicenda delle entrate che non sono state incorporate nel bilancio per l'ammontare di 34 miliardi di euro (operazione che andava fatta con una Nota di variazioni). Tra l'altro, c'è anche un errore formale perché l'emendamento al quale ci si riferisce è un altro, non c'entra niente. Quindi, se noi riteniamo la legge finanziaria e l'emendamento presentato un testo sacro, già quello starebbe a significare che c'è un errore formale di cui occorrerebbe tener conto. Signor Presidente, voglio concludere con una notazione: forse quello che ha detto con saggezza il presidente Andreotti non dovrebbe cadere. Forse, l'esercizio provvisorio per questa finanziaria, che non comprime la spesa ma mette molte tasse, sarebbe la soluzione migliore: lavorare per dodicesimi sarebbe la vera grande riforma di questa contabilità di Stato. Presidente, considero quella di stamattina un'occasione straordinaria per un parlamentare giovane di apprendere informazioni e notazioni originali e forse - devo dire - risolutive rispetto a questa dinamica della sessione di bilancio che unanimemente viene giudicata ormai ingestibile. Non c'è alcuno di noi che ritenga questa procedura

regionale siciliana ha il rango di Parlamento - e consideravo la prassi che utilizzavamo in Regione per formare la legge finanziaria accidentata, inadeguata, qualche volta persino imbarazzante nella congerie di interventi confusi che trovavano spazio in quella legge.

In questo documento (che nessuno di noi ha potuto, per le capacità che abbiamo, osservare, non dico minuziosamente, ma neanche superficialmente, con la conseguenza di ciò che realmente viene disciplinato) vi sono dei punti di conflitto fortissimi sul terreno costituzionale. Mi collego all'intervento del senatore Pastore. È davvero inaccettabile che attraverso la legge finanziaria vengano modificati gli Statuti regionali. In un Paese che si misura sul processo di federalismo, si evidenzia una lesione fortissima del rapporto pattizio esistente tra Stato e livello regionale.

che il Governo sequestri la funzione legislativa del Parlamento con questa legge, ma non si può contestualmente anche ledere il sistema delle autonomie e violare rapporti pattizi di rango costituzionale. Presidente, ho ascoltato l'intervento del presidente Morando che ha riferito secondo verità

sentiti i componenti della Commissione e del Gruppo Alleanza Nazionale e registrato che si trattava di un mero errore materiale, ho autorizzato a dire che si inserissero le

si è deciso, mi sembra unanimemente, che la Commissione facesse lo sforzo, che ha fatto in maniera assolutamente seria e lodevole.

questione di inammissibilità di alcuni commi. Per assoluto rispetto e trasparenza nei confronti del Senato ricordo, a proposito degli errori materiali, che il ministro Chiti ieri ha segnalato due ulteriori errori materiali di testo che sono i seguenti: al comma 1119 le parole: «già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione», andrebbero sostituite con le seguenti: «già realizzati e operativi». Questo è il primo errore. Il secondo riguarda il comma 1018. Sempre per errore materiale,

recita: «Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione». Circa questo punto la proposta che il Governo ha avanzato e che è inserita nel testo recepisce un accordo scritto intercorso tra la Regione ed il Governo stesso.

legge costituzionale dove si dà la possibilità a una legge ordinaria di modificare lo Statuto in alcune sue parti, questa norma viene superata dalla modifica dell'articolo 116 che non dà deroghe particolari a nessuna Regione per poter modificare con legge ordinaria il proprio Statuto. Quindi, credo che la modifica della Costituzione avvenuta nel 2001 cancelli e impedisca l'utilizzo delle norme ordinarie.

Bolzano. Il testo fa riferimento ad una serie di fattispecie ed andrebbe sostituito con un emendamento migliorativo, che era stato depositato in Commissione.

quell'articolo sarebbe scoperto.

preannunciato la formulazione di queste norme nella legge finanziaria, ma ho visto che invece, successivamente alla definizione di questi provvedimenti, è stato avviato una sorta di confronto contenzioso, che non ha trovato soluzioni condivise. vorrei comprendere se, anche in questo caso, avete ritenuto di applicare una procedura rispettosa delle norme o se, invece, dobbiamo sospettare che vi sia un regime giuridico diverso e un sistema di relazioni diverse a seconda del colore politico delle amministrazioni regionali. Pertanto, la Sardegna, che ha la fortuna di avere un'interlocuzione politicamente

Camera dei deputati che le condizioni del nostro lavoro sono tali che mi hanno impedito di consultarli prima. Cercherò, dunque, di spiegare correttamente la situazione. Queste sono le prime due questioni.

Per quanto riguarda i due emendamenti riferiti

Presidente, confermo che la norma che si propone per l'approvazione nel disegno di legge finanziaria recepisce un accordo scritto che è stato stipulato tra il Governo e il Presidente della Regione Sardegna. Visto che è stato fatto cenno anche alla Regione

recepisce un accordo tra Governo e Regione Friuli-Venezia Giulia. È stato oggetto di un protocollo di intesa, il quale, se non erro, è anche espressamente citato nella norma in questione con riferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

intervengo solo per sapere, salvo ovviamente le correzioni formali che accade sempre che si debbano fare, se lei ritiene chiusa questa fase, in maniera che da questo momento in poi

ha deliberato a favore dell'intesa di cui ha parlato testé il Governo. Quindi la procedura prevista dalla legge è stata espletata compiutamente. finestra"). Ho detto che ho bisogno di un approfondimento; non è che se ascolto altri suggerimenti salto l'approfondimento. È uno, ce n'è bisogno.

sessione di lavoro. Abbiamo proceduto, se ho ben capito, nel seguente modo. La Commissione bilancio si è espressa, ancorché non con un voto, ma con un'evidenziazione di questioni; il Presidente del Senato le ha recepite ed ha invitato il Governo a modificare il suo emendamento, intendendosi intendendosi con ciò che l'emendamento modificato veniva accolto dalla Presidenza del Senato. Questo è l'*iter* complessivo dei lavori, che può servire anche come precedente per i futuri lavori. Se è così, c'è naturalmente la massima condivisione da parte della nostra parte politica. Questa precisazione ai fini delle regole che restano mi pare assolutamente adeguata. Ma il Governo si è già pronunciato qui sulle questioni; quindi siamo d'accordo. Io mi sono riservato di pronunciarmi su una

la richiesta del Governo, a seguito della lettera

ordinamentali, mi permetto di sottoporre a lei e al Governo una norma contenuta nel maxiemendamento che potrebbe forse presentare qualche profilo di rilevanza al riguardo. Mi riferisco al comma 1346 che modifica la decorrenza dei termini di prescrizione della responsabilità contabile.

discussione, che ho seguito con grande passione, essendo non solo la prima finanziaria del Governo Prodi, ma anche la prima che seguo personalmente. Ho seguito tutto il percorso, appassionante ma anche troppo complesso,

Questa finanziaria non capita in un momento ordinario e quindi non poteva essere una finanziaria ordinaria. Vi è una fase nel Paese, ma direi anche in Europa, di disorientamento, di scollamento sociale, di difficoltà nel trovare riferimenti valoriali certi, una fase in cui è facile quindi ritirarsi un po' nella difesa eccessiva dei diritti individuali e anche corporativi, perdendo di vista un disegno sociale più complessivo, fatto di relazioni di identità culturali e valoriali diverse che si confrontano e rispetto alle quali la politica è chiamata, attraverso gli strumenti che le sono dati, a dare indirizzi di sviluppo precisi. La finanziaria è uno di quegli gli strumenti di cui dispone la politica per cercare di indirizzare questa società un po' spersa. Rispetto a questo quadro di insieme, mobile e fluido, difficile anche da interpretare,

Certo, lo sviluppo era complesso, ma anche doveroso, perché non possiamo permetterci di rimanere indietro. Ma nell'agganciarci all'aumento del PIL, quindi nel garantire misure reali di sviluppo al Paese, l'obiettivo doveva essere anche quello della redistribuzione del reddito. Allora c'è stato un percorso, sicuramente tortuoso e complesso, ne ho spiegato anche il perché, un *work in progress*, un po' affannoso e talora contraddittorio, perché anche dentro un processo democratico e partecipato, molto vissuto sulla stampa nazionale, è facile che sorgano contraddizioni e, talora, ci siano momenti comunicativi sbagliati. E questo è capitato soprattutto all'inizio. Ma ritengo che alla fine la finanziaria sia molto equilibrata tra chi deve dare e chi deve ricevere. È una finanziaria che, tra chi deve dare e chi deve ricevere, riesce a garantire la via dello sviluppo al Paese. Ce ne dobbiamo far carico tutti. Questa finanziaria tocca un po' tutti. È una finanziaria che carica maggiormente dal punto di vista fiscale chi guadagna di più,

Certo, sul sistema delle riforme dobbiamo essere tutti più coraggiosi; sul sistema della riforma e del federalismo fiscale dobbiamo lavorare nel corso del prossimo anno. I primi germi innestati con la legge finanziaria devono crescere, creare davvero i presupposti per un riordino complessivo del sistema fiscale nel Paese, dove l'elemento federativo deve essere importante, senza perdere di vista il principio di sussidiarietà,

delle riforme: le riforme non sono un problema ideologico; non dobbiamo citare riforme né da una parte né dall'altra in modo ideologico. Non sono sicuramente un modo per allarmare il Paese, ma una strada per risolvere i problemi. Quindi, le «riforme agitate» e le liberalizzazioni citate in modo ideologico, non servono: esse devono essere calate nella concretezza del Paese perché è là che dobbiamo risolvere i problemi e creare le condizioni per far ripartire la competitività.

abbiamo necessità di rivedere il sistema di formazione del bilancio. L'ho seguito per la prima volta, come ho detto all'inizio, con difficoltà: mi è parso un meccanismo complicato. Se andiamo verso una semplificazione della legge di bilancio, pur con un meccanismo partecipato, penso che facciamo un lavoro utile al Parlamento ma al Paese tutto, per chiarezza e trasparenza.

che non sono mirati e calati dall'alto, ma devono essere tesi a raggiungere una meta che tutti noi ci poniamo, in modo responsabile, in una fase difficile, in due anni che sono davvero cruciali per il rilancio del Paese. Se siamo tutti in grado di capire davvero quello che questa finanziaria propone e che i sacrifici non sono mirati semplicemente al al soddisfacimento di bisogni personali ma ad un bisogno collettivo, penso che possiamo davvero avviarci tutti su un cammino complesso che l'Unione con questa finanziaria ha voluto iniziare, ma che darà frutti importanti a tutti e al nostro Paese.

mi appresto ad ascoltare dai colleghi che compongono la 5a Commissione tutte le valutazioni complessive su questo Documento. intendo approfondire per il poco tempo che ho a disposizione due temi che mi stanno particolarmente a cuore, sui quali è gravemente carente questa finanziaria: i temi della montagna e del turismo. La montagna ha goduto proprio questa settimana di un momento di particolare attualità e di attenzione: l'11 dicembre, dal 2003, è celebrata in tutto il mondo la Giornata internazionale della montagna, istituita nel 2003 per l'appunto dal Governo Berlusconi, poi fatta propria dalla FAO e dalle Nazioni Unite. Da allora in tutto il mondo, in questa giornata, si richiama l'attenzione dei governanti e dell'opinione pubblica sulla specificità della montagna, sulle particolari condizioni di vita e di lavoro in queste zone. Va detto che è un tema che dovrebbe interessare anche la maggior parte dei colleghi, se è vero che all'Intergruppo parlamentare «Amici della montagna» hanno aderito 200 circa tra senatori e deputati. Va detto ancora che la montagna è una porzione importante, non solo della nostra economia ma anche della società

interessanti e incoraggianti di riconoscenza per chi vive e lavora in montagna, ma ha anche speso qualche promessa piuttosto precisa per le iniziative e le necessità di cui la montagna ha bisogno, al fine di alimentare il suo sistema economico e sociale, difendere l'ambiente, favorire condizioni di vita e lavoro competitive con le altre zone limitrofe ai territori di montagna, comprese le città e soprattutto per combattere quello che rimane il male più insidioso, cioè l'esodo da questi territori. Un esodo che è ancor più insidioso e pericoloso se riguarda i giovani. Se i giovani partono dalle montagne con essi se ne vanno anche le migliori prospettive di sviluppo per il futuro e si apre la strada a un degrado che non è solo ambientale ma anche sociale. Ecco per fermare questo *trend*, che appare inarrestabile, soprattutto nelle zone più periferiche d'Italia e del mondo, occorrono delle risorse.

comma 1287 non vi sono risposte ma soltanto notizie poco o per niente incoraggianti per chi vive e lavora in montagna. Innanzi tutto il Fondo nazionale per la montagna, previsto dall'articolo 2 della legge n. 97 del 1994, viene finanziato con ridicoli 25 milioni di euro e soltanto per il 2007. Non c'è neanche una previsione per gli anni successivi. Voglio ricordare che è vero che in questo esercizio erano soltanto 20 i milioni di euro a fronte di una sessantina richiesti, ma vorrei anche ricordare che nel 2005 il Governo Berlusconi mise a disposizione 31 milioni di euro e nel 2003 furono ben 61 i milioni di euro a disposizione del Fondo per la montagna. In compenso si istituisce un ente in più; è vero che poi se ne abolisce uno ma intanto si istituisce l'Ente italiano montagna, finalizzato, dice la motivazione, al supporto alle politiche e allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani, esattamente ciò che faceva o ha fatto fino a oggi l'IMONT (Istituto nazionale della montagna), che viene così soppresso e tutti i quattro commi successivi sono, non dico sprecati, ma dedicati alle modalità per il passaggio del patrimonio, del personale delle competenze, soprattutto dei finanziamenti per questo nuovo ente italiano della montagna. Va detto che su queste mancate previsioni, su questa mancanza di attenzione di considerazione verso la montagna si è espressa in maniera molto critica l'Unione nazionale dei Comuni enti montani, l'UNCEM, che critica in modo particolare l'attacco che viene sferrato al ruolo storico e alla funzione delle comunità montane come enti sovracomunali capaci di diventare autentiche cabine di regia per iniziative strutturali, sociali e di azione a beneficio della gente di montagna. Proprio l'UNCEM aveva indicato almeno in 61 milioni di euro lo stanziamento minimale e limite per poter fare qualcosa a beneficio delle zone di montagna, invece i 25 milioni riconosciuti sono francamente insufficienti. Veniva richiesta dall'UNCEM anche una maggiore valorizzazione dell'esperienza delle comunità montane per utilizzare le risorse fiscali del territorio montano, come le tasse di scopo e le imposte di soggiorno, le comunità montane rischiano di diventare meramente enti di carattere strutturale. Con una modificazione di natura burocratica da questo esercizio il Fondo per la montagna

e di prodotto interno lordo. È inutile illustrare in questa sede l'importanza che ha il turismo nella formazione del PIL nazionale. Il secondo atto decisamente criticabile nei confronti del turismo è quello di interpretare la competenza primaria - che, è vero, risale alle Regioni - come un alibi per ridurre a proporzioni ridicole le disponibilità finanziarie del Governo centrale.

il sostegno - così è definito - del settore turistico con soli 10 milioni di euro; il comma 1232 stanzia 48 milioni per tre anni

bastare per adeguare l'offerta sui mercati internazionali, migliorare i servizi, potenziare le strutture, difendere la proprietà dei beni di uso turistico e quindi dare un po' di morale a coloro che hanno nel turismo la loro professione prioritaria ed esclusiva:

lo stesso stanziamento di denaro, circa 50 milioni di euro, che il Governo prevede di riservare per tutta Italia. sul turismo non possiamo più fare finta di nulla nei confronti di quanto ci indica l'Unione Europea che, è vero, è sempre stata miope e disinteressata, considerando il turismo competenza

una comunicazione della Commissione europea impone ai Paesi membri di aumentare la *partnership* nei confronti del turismo europeo, auspicando quindi maggiore competitività, maggior comunicazione verso verso i Paesi terzi, strumenti finanziari potenziati e, soprattutto, un sostegno più esplicito e diretto alle imprese. Collego al tema del turismo grave occasione mancata che rappresenta anche una forte mancanza di rispetto verso centinaia di migliaia di cittadini italiani che abitano nel grande comprensorio turistico del lago di Garda, un comprensorio che tutto il mondo ci invidia. Dalla comunità del Garda credo che sia stato inviato un emendamento a tutti coloro che vivono in quella zona, che chiedeva semplicemente di ottenere il monitoraggio e la riqualificazione delle acque del lago di Garda attraverso la tecnologia applicata dall'istituto ICRAM.

di migliaia di abitanti delle sponde del Trentino. del Veneto e della Lombardia, che hanno nel bacino del lago di Garda non solo il loro *habitat*, e quindi intendono difenderlo sul piano dell'inquinamento; ma la loro principale reddito. In conclusione, signor Presidente, montagna e turismo sono due settori fragili e vitali che attendono da sempre una parola convinta da parte dei Governi. Essi, ancora una volta e ancora di più

a compiere un *iter* parlamentare e democratico. Quindi, ancora una volta, si dimostra - checché se ne dica - che vi è una metà del Paese che cerca di prevaricare sull'altra metà, e lo fa con logiche da basso impero, perché quando si arriva a 1.365 commi si si crea quasi uno stato di invidia con l'Impero romano d'Oriente: Bisanzio, infatti, avrebbe fatto sicuramente meglio, in tempi più rapidi e con maggiore efficienza. Tra l'altro, i dati forniti recentemente circa l'andamento delle entrate mostrano con chiarezza che non ci sarebbe stato bisogno di una manovra così forte e depressiva

(tradotti nel vecchio conio si tratta di 1.500 miliardi di vecchie lire) distribuiti a pioggia agli amici e ad associazioni più o meno strane: andiamo dagli apicoltori alle associazioni giovanili, fino a varie fondazioni, magari di Parma o di Firenze (cose di questo genere). Si tratta di operazioni di cui credo che il contribuente italiano non sentisse assolutamente la necessità. Non ne sentiva la necessità chi deve pagare l'imposta sul reddito delle persone fisiche, che vedrà aggravato il suo onere tributario già a partire da 20.000 euro lordi all'anno (che significa poco più di 1.000 euro netti al mese) e non mi sembra un reddito da grande capitalista; non sentivano questa necessità tutti coloro - credo che sia la totalità della popolazione italiana - che usano bere per poter sopravvivere: l'attuale Governo infatti ha messo anche un'imposta straordinaria sull'acqua minerale, come se essa fosse un consumo di lusso; in realtà, date le condizioni dei nostri acquedotti, si tratta di un consumo necessario. Siamo tornati, signor Presidente, all'imposta sul macinato: complimenti, per essere un Governo progressista. manovra finanziaria non provvede al risanamento, tant'è vero che nell'aggiornamento del Patto di stabilità e della partecipazione italiana si prevede una forte manovra per il prossimo anno (ciò vuol dire che il risanamento per il corrente anno non c'è); non provvede allo sviluppo, perché la forte manovra, combinata al fatto che è praticamente e interamente costruita sulla leva fiscale, impedirà uno sviluppo serio della economia italiana; infine, non ha nessuna caratteristica redistributiva - checché se ne dica - e questo non lo sosteniamo solo noi: basta chiederlo agli operai di Mirafiori. Quindi, cari signori, la manovra finanziaria è fallita da tutti i punti di vista.

fiscale. Se fosse così - ribadisco -, bisogna preferire dei limiti oggettivi, invece no: si definiscono dei limiti soggettivi perché obiettivamente ci può essere qualcuno che non è in grado di pagare con il contante. Ma cosa fa il Governo? Demanda a se stesso un decreto nel quale verranno indicate le categorie di cittadini impediti, cioè i poveracci a differenza degli altri. Quindi, quando magari un protestato - ci sarà anche qualche protestato non decisamente delinquente - necessiterà dell'intervento dell'idraulico, l'idraulico andrà a casa sua e il protestato dirà: «Non posso pagare con un assegno o con una carta di credito e, siccome sono protestato, dovrò pagare in contanti». In questo modo, tutto il quartiere avrà notizia di questo fatto. le persone che si trovano in maggior difficoltà, anche morale, saranno costrette ad esporsi perché questo Governo ama definire delle tassonomie e inquadrare i cittadini in categorie. In sostanza, quello che ne esce con chiarezza è che il

Da questo allo Stato etico, cari signori, il passo è molto breve; da questo a dire che i cittadini sono di serie A o di serie B, a seconda che corrispondano ad un criterio etico o ad un altro, il passo è brevissimo ed è un passo che porta ad uno Stato totalitario. Spero che ciò non accada, ma non vorrei che questo sia uno di quei piccoli passi che portano verso Vede, signor Presidente, a volte più delle misure cattive, irrazionali e sbagliate, forse fanno premio le misure ridicole

si riconoscono dei contributi finanziari a chi rottama l'automobile, non ne compra una nuova e sottoscrive un abbonamento al tram sul presupposto che sia meno inquinante che usare una macchina. Allora, cari signori, se uno va a piedi inquina di più rispetto a chi probabilmente non ci avete pensato, come non avete pensato al fatto che gli assegni di famiglia vengono corrisposti a chi ha un figlio che è studente oppure apprendista e non a chi ha un figlio disoccupato. Ciò accade probabilmente perché lo stato di disoccupazione è uno stato più vantaggioso rispetto a quello di studente. La misura ridicola sulla rottamazione è la seguente. Avete detto che la rottamazione ha senso se si sostituisce la macchina con una di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubi perché, giustamente, i poveri devono andare con una macchina che sia piccola e possibilmente dannosa in caso di incidente, mentre è giusto che si tutelino con macchine con carrozzerie più robuste i ricchi. Questo fa parte del vostro modo di pensare, esattamente come fa parte del vostro modo di pensare

Il che configura il seguente esempio: nel caso in cui ho una famiglia composta da marito, moglie e quattro figli ho questo *benefit*, mentre nel caso in cui la famiglia è composta da marito, tre figli e moglie incinta questo *benefit* non l'ho più. O devo aspettare che la signora abbia la creatura, oppure - ripeto - non posso avere questo *benefit*. Ciò mi sembra, oltre che irrazionale, francamente ridicolo e credo che, quando si supera la soglia del ridicolo, ci si mette in condizioni tali da non rendersi neanche conto di come va il Paese. Questo è quello che è emerso con palmare evidenza nelle ultime manifestazioni popolari, nei sondaggi e nella sensibilità generale. Ritengo che lo scollamento tra Governo e Paese stia diventando incolmabile. Una sola preghiera: fermatevi finché siete in tempo.

con la legge finanziaria si conclude quello che può essere chiamato il triangolo di politica economica di questo Governo all'inizio di questa legislatura. Non uso a caso questa figura geometrica, ma descrivo i tre lati del triangolo: il cosiddetto decreto Visco-Bersani di luglio, il decreto che è stato varato dal Senato un paio di settimane fa e la vera e propria legge finanziaria. Questo triangolo mostra che in realtà esiste una maggioranza formale, magari risicata, in Parlamento, ma è molto chiaro che all'interno di essa esistono alcuni specifici azionisti di riferimento ed è altrettanto chiaro che il Governo risponde, non alla sua maggioranza, ma a questi specifici azionisti di riferimento. Questi azionisti di riferimento sono all'esterno del nostro Paese e all'interno del nostro Paese. Palesemente, gli azionisti all'esterno del nostro Paese collegati ovviamente con l'*establishment* economico-finanziario - direi addirittura finanziario ed economico - che domina l'Europa e che guida le linee di politica economica europee al solo obiettivo di garantire l'equilibrio finanziario in modo che i creditori siano salvaguardati, indipendentemente dagli effetti che questo produce sull'andamento reale dell'economia. Su questo mi basta riferirmi a ciò che è avvenuto dall'inizio dell'*iter* del disegno di legge finanziaria ad oggi. Abbiamo cominciato a discutere di legge finanziaria

una burocrazia autoreferente decide, per esempio, di aumentare i tassi di interesse per un'atavica ed ancestrale paura dell'inflazione (che, chiaramente, risale nella storia alla Repubblica di Weimar, ma che non ha però alcuna possibilità di riscontrarsi nel presente e nel futuro) e, di fatto, questi dieci centesimi di apprezzamento ulteriore dell'euro azzerano completamente qualunque sforzo di qualunque Governo di qualunque politica economica all'interno dei Paesi aderenti all'area euro. Non si è levata mezza parola da parte del Governo italiano, come *partner* importante dell'Unione Europea, a discutere questo aspetto, non dico a contrastarlo ma a sollevare qualche dubbio. Francamente gli azionisti di riferimento interni

E allora, chiarito il punto politico che questa maggioranza non risponde alla propria maggioranza ma soltanto ad alcuni azionisti di maggioranza di riferimento, esterni ed interni, veniamo alla manovra.

la conclusione è che sul piano macroeconomico questa è la più grande operazione di puro potere di accentramento delle risorse e dei poteri nel Governo centrale che mai sia avvenuta nella storia della Repubblica italiana. È il più forte spostamento di peso a favore dello Stato sottratto ai cittadini, ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese, sia sul fronte economico che su quello delle libertà civili. Sul piano microeconomico - e basta leggere attentamente, cosa che abbiamo fatto nel corso della notte, i 1.365 commi del maxiemendamento

con le quali il Governo corre dietro - o meglio si fa correre dietro - addirittura inserendo nel testo consegnato una colonna in ogni pagina, per risalire con nome e cognome a chi ha chiesto quell'emendamento e

ha chiesto ed ottenuto queste marchette attraverso i 1.365 commi. Ma l'aspetto sorprendente, che dimostra l'evidenza della presenza di azionisti di riferimento, che rende estraneo il singolo parlamentare della stessa maggioranza alle decisioni della legge finanziaria, che rende estranei

si leggono più nomi di dirigenti di Ministeri e di associazioni di categoria. Pur non risultando in modo esplicito si possono intuire i nomi di singole specifiche imprese, di singoli specifici settori. Ebbene, quest'operazione macroeconomica di spostamento di potere, confusa nel polverone microeconomico

è stata poi supportata ed è sinergica - considerato che il polverone serve a coprire la verità vera di questa manovra - allo spostamento di potere. E chi è che ha le leve del potere dentro questo Governo? È stata ovviamente condita da palesi falsi in comunicazione sociale e da due palesi falsi in bilancio e allora si spiega l'*iter*. Una prima finanziaria varata dal Governo nel Consiglio dei ministri del 28 settembre scorso, cambiata tre giorni dopo quando il Ministro dell'economia e delle finanze presenta insieme al Presidente del Consiglio a Milano in conferenza stampa un altro numero,

ma come il vecchio Gattopardo la finanziaria è stata cambiata quattro volte perché nulla cambi delle colonne portanti di questa finanziaria.

della Costituzione - questa finanziaria determina un aumento di entrate (tasse, per parlare chiaro, nelle varie versioni) pari a 35 miliardi di euro per coprire un aumento di spesa pubblica corrente. Nella tabella ufficiale, o semiufficiale, allegata è riportato un aumento di spesa pubblica corrente di 25 miliardi di euro, concentrati nei portafogli di 12 Ministri. Questo è il flusso che si determina. Escono soldi dai portafogli delle famiglie e delle imprese ed entrano in quelli dei Ministri, che poi, a loro discrezione, a pioggia, nei vari commi

e mostra a ciascuno la possibilità di accaparrarsi un sacchettino di pane grattuggiato. Questa è la politica economica del Governo Prodi: 35 miliardi, con questa finanziaria, per consentire aumenti di spesa pubblica corrente dichiarati dal Governo. A questi si aggiunga

il falso in bilancio dimostrato dallo stesso Governo pochi giorni fa, relativo all'andamento delle entrate nel 2006;

Però, purtroppo, i numeri sono numeri e quella verità dice che al 30 novembre 2006 vi sono stati 34 miliardi di entrate in più rispetto al 2005; lo stesso vice ministro Visco correttamente ha detto che a fine dicembre saranno qualche altro miliardo in più. Note interne delle varie amministrazioni indicano questo «di più» in circa 37-38 miliardi, ma il falso non sta soltanto nel totale, che finalmente il Governo ha reso noto al Paese, bensì nella sua composizione perché da quella stessa tabella gli incrementi di IRPEF su lavoro autonomo e su lavoro dipendente, gli incrementi di contributi sociali su lavoro autonomo e su lavoro dipendente dimostrano il grande e positivo effetto della legge Biagi. Saranno lavori flessibili, saranno lavori precari, ma non sono lavori neri e quindi pagano IRPEF e contributi sociali. Questi sono incrementi di entrate strutturali e permanenti. L'incremento dell'IVA, ovviamente agganciato alla ripresa economica, è strutturale e permanente, a meno che non si abbia il retropensiero - come posso come posso dimostrare e ho tentato di fare in altre occasioni - che poiché questa finanziaria ammazza la crescita, di conseguenza ucciderà anche l'incremento delle entrate pubbliche. Il falso in bilancio consiste nell'aver dichiarato 38 miliardi di euro di entrate in più, nell'aver constatato che nella tabella, secondo le varie voci, almeno 25 miliardi di euro - voglio essere generoso generoso - sono strutturali e permanenti e andavano messi nel bilancio di previsione 2007 con una Nota di variazioni. Il Governo ha rifiutato e continua a dichiarare che vi metterà solo cinque miliardi. Quindi, fate attenzione: potete fare tutti i polveroni che volete, facendo credere che mettete l'imposta di soggiorno e poi la togliete, che mettete la tassa di successione e poi l'aggiustate. Non confondete, però, gli occhi degli italiani con questi polveroni, perché è chiaro che sta portando a casa di 12 ministri 55 miliardi di euro, 35 con la finanziaria e 20 con quelli, chiusi nel cassetto, che non avete voluto correttamente inserire nella Nota di variazione al bilancio. Questo, a mio parere, è un falso in bilancio; avevo presentato pure una questione sospensiva. Ho anche aggiunto che queste tabelle, in altre occasioni, con altri Presidenti della Repubblica, non sarebbero pervenute nelle Aule parlamentari in tali condizioni.

Il presidente Prodi forse non ha letto le previsioni del Ministro dell'economia e delle finanze e non solo quelle di importanti

ha scritto, e poi confermato in Commissione, che l'effetto di questa manovra è depressivo. Vi è una differenza,

la falsa comunicazione sociale che questo Governo ha fatto e continua fare quando afferma che la manovra mira ad ottenere sviluppo economico, equità sociale e risanamento finanziario. Vengo ora proprio al risanamento finanziario.

li avrei perseguiti, il centro‑destra li avrebbe perseguiti, andando a prendere le risorse con il contenimento della spesa corrente, non con l'aumento delle tasse. Anche aumentando le tasse, il centro‑destra avrebbe avuto in mente un'idea di progetto strategico. Così non in questo maxiemendamento. Chiudo rapidamente, citando alcune cose che smascherano gli azionisti di riferimento e per qualche aspetto - come ha già detto il collega Vegas - assumono un carattere francamente ridicolo ed irrisorio. Prendo atto che la sinistra, usata per tanti anni ad essere - come si diceva - *politically* *correct*, oggi è diventata «*hypocritically*

Il comma 53 - laddove modificate la successione per i fratelli, eccetera - vale a partire dai decessi avvenuti dopo il 3 ottobre 2006. Forse pensate

i commi, palesemente con nome cognome (lo ha già detto il collega Vegas), sulle SIIQ (azionisti di riferimento).

che il TFR presso le imprese non rappresenta un debito delle imprese; anche in questo caso, il povero Fra Luca Pacioli si rivolta nella tomba sulle regole normali della contabilità. *(Applausi

alcune considerazioni sull'aspetto dello sviluppo. È stato detto che questa manovra, così grossa nelle dimensioni, è anche orientata a creare lo sviluppo dell'economia del nostro Paese. Allora, la domanda che ci dobbiamo porre è molto semplice: dopo questa finanziaria l'Italia crescerà di più? Sarà più competitiva?

notevole e forte della pressione fiscale. Credo di non dover perder tempo nel dire che nessuna teoria economica e nessuna osservazione empirica può dimostrare che, aumentando le tasse, si aumenta la capacità di sviluppo e di competitività di un sistema Paese. Quindi, il primo motivo deve individuarsi nel livello ormai altissimo della pressione fiscale nel nostro Paese, a seguito delle varie manovre del Governo Prodi.

Il cuneo fiscale è semplicemente un aiuto finanziario *una tantum* alle imprese, su un fronte che non è determinante per la competitività del nostro Paese. Abbiamo un *gap* di costo del lavoro di 1 a 10, 1 a 50, 1 a 100 i nostri maggiori concorrenti. Un intervento così limitato sul cuneo fiscale certamente non migliora la nostra posizione competitiva. quanto riguarda poi la ricerca e l'innovazione, che sono i veri motori di competitività e di crescita di una moderna economia, per farla breve, visto il tempo che ho a disposizione, dico che questa finanziaria riduce e non aumenta, come invece qualcuno ha affermato, le risorse finanziarie nella filiera della ricerca e dell'innovazione.

la competitività e lo sviluppo del Paese dipendono anche dall'efficienza della produttività della pubblica amministrazione. E allora sfido chiunque a leggere le 385 pagine di questo maxiemendamento e a trovare una sola

per quanto riguarda la pubblica amministrazione ed è prevista una miseria - sottolineo: una miseria - di soli 10 milioni di euro per lo sviluppo di iniziative relative alla società dell'informazione.

non si può impostare oggi una politica a sostegno dell'innovazione industriale, e quindi della competitività delle imprese, dando allo Stato il compito di scegliere dove investire. Si tratta davvero di qualcosa ormai

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora poche ore e domani sera dovrebbe essere approvata la più modificata, la più contestata, la più avversata legge finanziaria degli ultimi anni. A questo punto ci saremmo aspettati, se non dal Ministro dell'economia, al quale l'alto incarico ministeriale, invece di aggiungere, ha invece sicuramente tolto gran parte del prestigio e della credibilità, quanto meno dal Presidente del Consiglio un commento prudente e misurato sulla natura e sugli effetti della manovra. Al contrario il *Premier*, probabilmente non pago dei fischi e delle contestazioni massicciamente accumulate negli ultimi giorni, sadomasochisticamente ha continuato a difendere questa sciagurata manovra finanziaria attribuendo, si guardi un po', le reazioni delle categorie e dell'opinione pubblica a un semplice difetto di comunicazione e ad alcuni errori tattici. Converrà però il Presidente del Consiglio che una opposizione che ha dimostrato, anche in questo ramo del Parlamento, la propria cultura politica, la propria saggezza politica, un proprio senso di responsabilità politico, non poteva accettare supinamente questa giustificazione, perché, se di errori si deve parlare, allora si deve parlare non solo di errori tattici, ma anche di errori strategici. Se al presidente Prodi, impegnatissimo in questi giorni nell'eccessivo scambio di affettuosità con il *premier* israeliano Olmert, sfugge qualche particolare, è nostro dovere, dovere di questa opposizione, dovere di Alleanza Nazionale, ricordargli che cos'è e che cosa rappresenta questa legge finanziaria. È una legge finanziaria condizionata da fortissimi contenuti ideologici, tant'è che rimarrà negli annali la vostra teoria secondo la quale anche i ricchi dovrebbero piangere. In sostanza una riedizione di quella lotta di classe targata anni Sessanta e Settanta, che tanti drammi e tanti lutti procurò al nostro Paese. È una legge finanziaria che sancisce il vostro fallimento rispetto ai tre aspetti principali che avrebbero dovuto invece caratterizzare una positiva politica economica: incidere sui parametri del debito pubblico, conseguire l'obiettivo di un'equa redistribuzione del reddito, raccogliere almeno il consenso delle categorie sociali più deboli. Nulla di tutto questo, dobbiamo dirlo con chiarezza, è avvenuto. Nonostante una congiuntura economica internazionale sicuramente più favorevole rispetto a quella con la quale dovette confrontarsi il centro-destra; nonostante i segnali di ripresa della nostra economia, già avvertitisi negli ultimi mesi del Governo Berlusconi; nonostante il *boom* delle entrate tributarie, che impudentemente avete cercato di accreditare alla vostra politica fiscale, quando è noto a tutti che queste entrate straordinarie costituiscono la naturale conseguenza della politica fiscale del centro-destra, una politica fiscale caratterizzata dal ribaltamento di un vecchio e devastante schema, che è il vostro schema: il fisco come nemico del cittadino; nonostante tutto questo, possiamo dire che col centro-destra questo schema è diventato un'altra cosa: fisco e cittadino insieme per sostenere il sistema Paese grazie ad una pressione fiscale equa e sopportabile. Una manovra, quindi, che non esitiamo a definire depressiva, repressiva, inopportuna e punitiva. Depressiva, perché incide negativamente sul sistema delle imprese che, nel saldo tra presunti benefici derivanti dall'introduzione del cuneo fiscale da un lato e aumento degli oneri sociali, della fiscalità generale e locale e introduzione del TFR dall'altro, cederà altri margini di competitività. Dopo questa legge finanziaria le imprese italiane saranno sempre meno competitive e soprattutto sarà destrutturato il sistema di quelle piccole e medie imprese che sono state ignobilmente trascurate da questo Governo. Repressiva, perché introduce un sistema da stato di polizia: *ticket* ospedalieri, tracciabilità dei pagamenti, violazione permanente dello Statuto del contribuente. Avete tentato anche di violare il principio di irretroattività delle norme fiscali, mettendovi sotto i piedi e calpestando i principi fondamentali della Costituzione e del diritto. Inopportuna, in quanto ancora non avete spiegato i motivi per i quali non siete stati consequenziali a quanto dichiarato qualche giorno fa a Forlì dal Ministro dell'economia.

le risorse eccedenti 15 miliardi sono state utilizzate per soddisfare la voracità dei *partner*, dei cespugli, di tutta quella miriade di piccoli soggetti politici che oggi costituiscono l'ossatura del Presidente del Consiglio, visto che non possono costituirla i partiti maggiori. E consapevoli di questa situazione questi piccoli partiti lo ricattano. Ma questo è un gioco scoperto. Lo hanno capito le categorie, i lavoratori di Mirafiori, i tassisti che ieri con molta delicatezza hanno manifestato al presidente Prodi tutto il loro «affetto» attraverso una salva di fischi non aventi una natura americana! Lo hanno capito soprattutto i due milioni di cittadini che qualche giorno fa hanno invaso spontaneamente e pacificamente Piazza San Giovanni con un messaggio ed un auspicio: questa finanziaria sia non solo l'ultima del Governo Prodi, ma anche della sua maggioranza. Signor Presidente, intervengo sulla parte che riguarda più da vicino il comparto agricolo ed agroalimentare di questa manovra finanziaria, sia per quanto riguarda il risultato del lavoro svolto dalla Camera dei deputati (quindi la finanziaria che abbiamo ricevuto al Senato), sia per quanto riguarda le modifiche apportate attraverso il maxiemendamento. il maxiemendamento. Si tratta di una finanziaria sicuramente importante e molto positiva per l'agricoltura, a testimonianza di quello che avevamo detto in campagna elettorale, cioè che questo Governo avrebbe avuto rispetto al mondo agricolo ed agroalimentare una attenzione particolare identificandolo come uno dei settori su cui puntare per il rilancio del nostro sistema Paese, essendo uno dei settori che hanno maggiore valenza non solo economica ma anche sociale ed ambientale. Ebbene, queste affermazioni nella campagna elettorale, nel programma dell'Unione sono state ampiamente corrisposte da un'attenzione particolare e da norme ben specifiche sul comparto agricolo. Avevamo detto nel programma per l'agricoltura dell'Unione che due sono i temi che l'agricoltura italiana deve affrontare: uno è quello della competitività delle imprese agricole per fronteggiare la concorrenza dei mercati globalizzati; l'altro è quello di una attenzione particolare agli aspetti della commercializzazione dei prodotti agricoli. agricoli. Se noi tutti siamo convinti che l'agricoltura italiana debba e possa essere solo un'agricoltura di qualità, un'agricoltura con forte radicamento nei nei propri territori per quanto riguarda le produzioni tipiche e la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, di cui è ricchissimo il nostro Paese per cui è ammirato in tutto il mondo (ricordiamo che il *made in Italy*, ancora prima che moda e automobili di lusso, è *made in italy* agroalimentare); se se è vero che dobbiamo improntare le strategie di sviluppo dell'agricoltura ad una agricoltura di qualità, è anche vero che questa qualità deve essere pagata, remunerata ai produttori agricoli perché fino a quando ci riempiremo la bocca della parola qualità, ma non riusciremo a farla valorizzare sul mercato interno, ma soprattutto sui mercati internazionali per quello che vale e per quanto è apprezzata nel mondo, le nostre imprese agricoli chiuderanno. Allora, già alla Camera vi erano numerose iniziative legislative nell'ambito della manovra finanziaria che andavano nel senso di un aumento della competitività delle imprese e di una messa a disposizione di strumenti più efficaci per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Innanzitutto, vi è il riferimento al comparto agricolo per quanto riguarda il cuneo fiscale, sebbene - lo abbiamo detto anche in Commissione agricoltura la riduzione del cuneo fiscale per gli operai a tempo indeterminato non riguardi in misura importante l'agricoltura, nel momento in cui più dell'85 percento dei dipendenti agricoli sono dipendenti a tempo determinato. rimane un forte impulso dal punto di vista della competitività delle imprese per quanto riguarda il costo del lavoro e quindi questa è sicuramente un'iniziativa positiva.

extracomunitaria in agricoltura. Se vogliamo parlare di un'agricoltura di qualità non possiamo parlare di un lavoro di qualità in agricoltura. Quindi, l'obbligatorietà del Documento unico di regolarità contributiva, il DURC, per poter percepire contributi comunitari, come pure la comunicazione telematica all'INPS dei rapporti di lavoro vanno nel senso di una maggiore tutela del lavoro, ma soprattutto di un lavoro di maggior qualità. maggior qualità. Ci sono altre norme importanti per quanto riguarda la competitività delle imprese. Innanzitutto, il credito di imposta, che poi per il Sud, con una norma inserita nel maxiemendamento, è stato

l'istituzione di un fondo per favorire la penetrazione commerciale all'estero e l'adozione di marchi consortili dei prodotti*made in Italy.* Abbiamo poi un'importante norma sulle vendite dirette

160.000 euro. Vi sono poi norme che riguardano gli strumenti, le forme societarie.

Al Senato si è andati ulteriormente avanti su questo tema, introducendo la possibilità che società agricole possano occuparsi anche semplicemente della trasformazione, commercializzazione e promozione dei propri prodotti, quindi indipendentemente dalla produzione stessa. È una norma molto importante che fornisce al comparto agricolo uno strumento molto importante per quanto riguarda la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

Questa norma è stata recuperata al Senato nel maxiemendamento, con una dotazione finanziaria non irrilevante, di 10 milioni di euro, che si aggiungono ai 5 milioni di euro che erano stati stanziati dal Governo di centro-destra e dal Ministero guidato È un'attenzione importante che vogliamo dare all'agricoltura biologica, che non consideriamo un settore residuale ma un'opzione importante per la nostra agricoltura e per un modello di agricoltura che l'Unione vuole incentivare in grande

al Senato si è riusciti ad inserire nel maxiemendamento alcune norme sui biocarburanti che mostrano particolare attenzione alla produzione di energia da parte del comparto agricolo.

prodotti dalle imprese agricole, che subiscono un trattamento di equiparazione alle altre produzioni di olio vegetale sempre da materia prima agricola.

nella considerazione che il terreno è un *input* produttivo classico dell'attività agricola e che, quindi, se c'era un trasferimento in successione dell'impresa, doveva essere comunque considerato in maniera differenziata dalla tassazione per i beni patrimoniali privati. Questo concetto è entrato nel maxiemendamento; naturalmente esso non concerne soltanto l'agricoltura, ma la riguarda

l'estensione alla cooperazione e alle imprese agricole delle agevolazioni fiscali sull'internazionalizzazione dei prodotti e la promozione del *made in Italy* agroalimentare, l'istituzione delle società agricole per la trasformazione e la commercializzazione del prodotto, il credito d'imposta per la certificazione di qualità, secondo cui le imprese che aderiscono a progetti di certificazione di qualità possono ricevere crediti

Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli senatori, ci sono mille motivi per opporsi a questa finanziaria, quasi quanti sono i commi del maxiemendamento. In realtà, ce ne sarebbero mille e uno, dove l'ultimo motivo per dichiararsi contrari a questa finanziaria sta proprio nel maxiemendamento, e per le procedure con cui è stato presentato, non ultimi i tempi che non hanno consentito a tanto di noi di prendere una visione reale del testo.

Che non ci fosse il rigore lo avevamo capito dall'inizio, non fosse altro che leggendo gli attestati degli istituti internazionali di certificazione, che hanno immediatamente declassato il debito del nostro Paese: abbiamo letto l'ultima attestazione proprio ieri. Le motivazioni sono semplici: non ci sono tagli strutturali, non c'è un accenno a quel processo di liberalizzazione di cui si parla tanto nei giornali e nei convegni, non c'è una riga sui temi come le pensioni e la pubblica amministrazione, che sono nervi scoperti di questa maggioranza. Si procede attraverso l'aumento della pressione fiscale; in realtà, tutti sappiamo

sono state toccate tutte le categorie sociali, ma in particolar modo le categorie produttive - citando il senatore Curto - forse facendo piangere i ricchi, ma sicuramente

ma conseguentemente per l'intero Paese. Credo che non sia assurdo sostenere che tale manovra fiscale tende a congelare le attuali strutture di reddito e le di reddito e le attuali articolazioni sociali del nostro Paese; in questo senso la considero una manovra conservatrice. Detto questo, il Mezzogiorno e le aree deboli

(semmai lo consegnerò nel testo scritto che lascerò alla Presidenza, perché è una materia di mio particolare interesse), ma le risorse per il Mezzogiorno sono inferiori a quelle allocate dai precedenti Governo e sono molto inferiori rispetto a quelle promesse.

storica, culturale, geografica, ambientale e insediativa, che chiede di opporsi a questa finanziaria che va contro i suoi interessi e i suoi bisogni. Non sarei coerente con me stesso se non mettessi i bisogni e le attese della mia comunità regionale - sto parlando della Sardegna - al centro del mio ragionamento. Non sarei coerente con me stesso se non dicessi che questa finanziaria

cancella due dei pilastri fondamentali sui quali si sono rette tutte le intese pattizie tra Stato e Regione: la sanità e i trasporti.

dare una risposta a una sacrosanta battaglia della Sardegna sulle entrate, portata avanti da tutti Governi, di centro-sinistra e di centro-destra. Questa mattina si

ma non è altrettanto lecito sul piano politico, soprattutto perché il Consiglio regionale, che ha dato il proprio assenso formale, l'ha fatto a cose

del saldo del debito sulle entrate pregresse e non pagate negli scorsi anni e concede altresì alla Sardegna un nuovo calcolo dell'imposta IVA a partire dal 2010. Per contro,

Non mi soffermo, perché è stato già fatto, sul presunto equilibrio dell'accordo tra il Ministro dell'economia e il nostro Presidente della Regione tra le nuove entrate e la spesa sanitaria, se non per dire che questa va a svantaggio della nostra Regione, se appena si tiene conto degli incrementi percentuali, dovuti all'inflazione, del costo per la sanità e se si tiene conto delle nuove risorse per il Sistema sanitario nazionale di cui la Sardegna non potrà godere.

Per quanto riguarda il sistema dei trasporti, in particolare il trasporto locale, mancherà la partecipazione dello Stato a gestire due strumenti di trasporto, due aziende come le Ferrovie meridionali e le Ferrovie della Sardegna, che assicurano l'accessibilità in aree marginali e - perché non dirlo? - emarginate della nostra Regione in qualche maniera sostengono un sistema di trasporti locali che non voglio definire da Terzo mondo, ma è sicuramente non moderno, non efficiente, non europeo, basato su un sistema ferroviario che fa pena e su un sistema stradale in cui i livelli di servizio sono i più bassi fra tutte le Regioni italiane e la cui estensione, rispetto alla superficie territoriale, è di gran lunga la più bassa.

attraverso risorse pubbliche. Queste risorse pubbliche d'ora in poi saranno a carico della Regione. Lo stesso capiterà per il trasporto marittimo. Fra qualche anno considerata la proroga data alla convenzione tra lo Stato e la Tirrenia - alcune rotte, solo alcune ma importantissime che non si reggono sul mercato, dovranno essere messe sotto protezione. Anche per questi motivi, Anche per questi motivi, ma vorrei dire soprattutto per questi motivi, il mio voto sulla finanziaria sarà contrario.

Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, questa finanziaria almeno un merito lo ha avuto: chiarire che l'anima riformista della maggioranza è costretta a sottostare al *diktat* della sinistra radicale e al legame incestuoso con il sindacato confederale, in particolare del settore del pubblico impiego. Oggi, infatti, il vero potere di pressione è nelle mani del sindacato, della CGIL in particolare, che rappresenta i pubblici dipendenti. Lo è per la maggior disponibilità di risorse, lo è per il presunto potere di condizionare le scelte elettorali dei suoi iscritti. Per questo non sorprendono i fischi che hanno salutato la visita di Epifani a Mirafiori. Essi hanno commentato, in forma sonora, la volontà del sindacato di ignorare le trasformazioni sociali in atto, anche al prezzo di chiudere gli occhi e tapparsi le orecchie al cospetto di nuovi bisogni e di inedite debolezze. I pubblici dipendenti, assieme ad alcune categorie di pensionati, sono divenuti il vero blocco sociale di riferimento dell'attuale maggioranza. Non casualmente, i lavoratori della pubblica amministrazione rappresentano l'unica categoria ad aver ottenuto riconoscimento in questa manovra finanziaria attraverso il trasferimento di ingenti risorse (quasi un quinto dell'intera manovra per il prossimo biennio). Se servisse un'ulteriore conferma di ciò, basti ricordare come i sindacati hanno preteso, e nel giro di qualche giorno ottenuto, una modifica normativa che sostanzialmente smantella il sistema dei controlli. Per completare l'opera, hanno anche preteso la rimozione dei vertici dell'ARAN. Fatti saltare i controlli, garantita un'ARAN «amica», il rischio concreto è che i contratti collettivi del pubblico impiego finiscano per trasformarsi in contratti unilateralmente scritti dai sindacati in splendida solitudine. Nei giorni scorsi l'offensiva sindacale si è allargata fino a comprendere anche la Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici e non è mancato nemmeno il tentativo di decimare la dirigenza della Ragioneria generale dello Stato. Lo scorso 12 novembre, in un articolo pubblicato sulle pagine de «l'Unità», il professor Paolo Prodi invitava ad una comune riflessione sull'anomalia del ruolo del sindacato in Italia, denunciando come i gangli del potere siano oggi presidiati da uomini del sindacato, e sulla necessità di reintrodurre, nel rispetto delle funzioni, una netta separazione tra sindacalismo e politica. Ministro Padoa-Schioppa, siamo prossimi al Natale. Per la quiete delle famiglie s'incarichi lei di spiegare al fratello del Presidente del Consiglio che non è possibile, almeno finché questo Governo resterà in carica. Il sindacato, infatti, pretende di scegliere i propri interlocutori istituzionali: una situazione che gli economisti definiscono *capture*, ovvero la cattura del regolatore da parte degli interessi regolati. E «Prodi *le* *petit*» non potrà proprio dare soddisfazione al fratello maggiore, perché, dopo la *liaison* ancora insoluta tra politica e magistratura, quella con il sindacato rappresenta l'altro conflitto d'interesse della sinistra italiana! Anche per questa ragione non sortiranno effetti le richieste del ministro Rutelli che, in cambio del presunto rigore offerto in termini di finanza pubblica, si aspetta il consenso dei sindacati su un'operazione di liberalizzazioni e rilancio economico. Ministro Rutelli, se fosse questo l'intento del vostro azionista di riferimento, non sareste stati costretti ad una manovra finanziaria che agli inauditi sacrifici richiesti non ha fatto corrispondere alcun taglio della spesa strutturale, né riforme che possano aiutare il rilancio dell'economia, né l'ammodernamento delle infrastrutture del Paese. Questa è la contraddizione di fondo della quale rimarrete vittime: avete voluto fare una manovra finanziaria di lacrime e sangue all'inizio della legislatura contando sul tempo di sedimentazione del giudizio che i meccanismi della democrazia rappresentativa vi consente. Ma i vincoli strutturali che l'azionista di riferimento vi ha posto e vi continuerà a porre, faranno sì che nessun alleggerimento della pressione, nessuna riforma di struttura, nessuna opera d'ammodernamento seguirà questo rito sacrificale collettivo che state imponendo al Paese. E, alla fine, il tempo trascorso giocherà contro di voi rendendo ancora più catastrofico il giudizio degli italiani sul vostro operato. Ministro Rutelli, lei sa quanto me che una seria politica di sviluppo in termini di competitività sarà possibile solo se si interverrà sui meccanismi che governano il funzionamento della pubblica amministrazione. Le soluzioni, però, possono essere anche diametralmente opposte e questa manovra finanziaria lo dimostra. Noi siamo per un controllo della spesa accompagnato da un autentico riconoscimento per quei lavoratori pubblici realmente capaci e meritevoli. Voi, invece, state assecondando il sindacato nel concedere aumenti retributivi e premi di produttività a pioggia. Noi immaginiamo una dirigenza responsabilizzata e incentivata in base alle *performance* delle amministrazioni di riferimento. Voi state mortificando la dirigenza sottoponendola a continui tentativi di *spoils* *system*. Noi siamo per il rigore nei controlli di compatibilità economica dei contratti. Voi li volete affidare nelle mani dei soli sindacati. Noi siamo contro l'iniqua differenziazione delle retribuzioni nel settore privato e in quello pubblico. Voi non vi scandalizzate che il pubblico si ponga alla stregua di un settore protetto, al riparo di ogni seppur minima influenza delle leggi di mercato. Noi siamo per la trasparenza delle prerogative sindacali nel pubblico impiego. Voi continuate a porre il prezzo di distacchi e privilegi sindacali sulle spalle del contribuente. Se si applicassero i vostri criteri nel settore privato, la quasi totalità delle imprese oggi sarebbe già fallita. Per un residuo di mentalità comunista, per tanti di voi sarebbe un auspicio. Per il Paese una rovina che noi cercheremo di non farvi realizzare.

di dire qualcosa sulla mia terra di Sicilia. Ho percepito nello sguardo degli ulivisti una falsa contentezza rispetto agli investimenti che questo Governo ha previsto per la Sicilia.

Sicilia. Fra qualche giorno il dottor Bondi consegnerà i documenti al tribunale per dichiarare il fallimento dell'ultimo residuato industriale della Parmalat in Sicilia. Qualche giorno fa il dottor

della piattaforma logistica per la realizzazione degli interporti in Sicilia. Quindi, la Sicilia è espropriata da tutto e su tutto. Niente occupazione, niente ponte, niente termovalorizzatori, niente piattaforma logistica, niente di tutto ciò, né tanto meno

finanziaria)** Le nuove norme in materia ambientale inserite nel maxiemendamento rendono ancora più confusa, frammentaria e priva di un disegno strategico la politica dell'ambiente . Più che un corpo omogeneo, il maxiemendamento propone ancor di più del testo licenziato dalla Camera, un insieme disordinato di interventi *spot*, spesso contraddittori tra di loro, di misure inutilmente penalizzanti che fanno ben poco per incidere in maniera concreta e sistematica in un settore, come quello dell'ambiente, primario per lo sviluppo del Paese e la vita dei cittadini. Il dato più preoccupante di questa legge finanziaria è comunque costituito dalla evidente assenza di una strategia per la politica ambientale. Tale evidente assenza di strategia risulta ancor più criticabile se si considera che, nella scorsa legislatura, la conduzione del Dicastero dell'ambiente e delle politiche ambientali è stata contraddistinta invece dal fermo e coerente perseguimento di precisi e meditati obiettivi da parte dell'allora ministro obiettivi chiaramente indicati all'atto della presentazione del disegno di legge delega ambientale, sulla base del quale è stato poi adottato il decreto legislativo n. 152 del 2006, il cosiddetto Codice ambientale. Con quest'ultimo il precedente titolare del Ministero dell'ambiente ha saputo fare ciò che nessuno, in precedenza, era stato capace di realizzare e cioè la raccolta e l'aggiornamento, in un *corpus* organico, di tutta la normativa ambientale sulla base di finalità e di princìpi organici, esaminati preventivamente ed adeguatamente meditati dal Parlamento. Un esempio della mancanza di un disegno organico di questa finanziaria sono le norme che riguardano i rifiuti. Da una parte si attua una politica di retroguardia (comma 184), rimandando *sine* *die* l'entrata a regime della tariffa sui rifiuti, uno dei pilastri per il perseguimento di una politica di riduzione di produzione dei rifiuti, dall'altra si fanno salti in avanti del tutto velleitari difficilmente realizzabili, come le disposizioni contenute nel comma 1111, che prevedono una raccolta differenziata entro fine 2007 di almeno il 40 per cento, che deve salire fino al 60 per cento entro il 2011, pena il commissariamento. Con una misura del genere si vedrebbe praticamente tutta l'Italia commissariata per i rifiuti, visto che la media della raccolta differenziata in Italia è del 23 per cento e l'unica Regione al di sopra del 40 per cento è solo la Lombardia. Sempre per quanto riguarda i rifiuti, il comma 186 proroga il conferimento in discarica dei rifiuti non trattati, ma non proroga il termine per i rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kilojaul/kg, che quindi non potrebbero essere più smaltiti in discarica dal 1° gennaio 2007. Si tratta ad esempio di rifiuti come il *fluff* (le parti di tessuto e di plastica delle vetture non recuperabili) che non troverebbero più una destinazione visto che la loro destinazione naturale, gli inceneritori, non si sono costruiti né si costruiranno. E questo è tanto più grave visto il vasto programma di rottamazione delle auto previsto

Presidente, nella giornata di ieri, discutendo sulle questioni di bilancio, alcuni senatori dell'opposizione (Grillo, Cicolani e Ferrara), manifestando una diversa conoscenza della materia di cui stavano discutendo (in particolare mi è parsa ostica la materia dalle osservazioni fatte dal senatore Ferrara), hanno in pratica demolito la politica infrastrutturale di questa finanziaria e hanno, invece, eretto un monumento al quinquennio del centro-destra che si è aperto con quella monumentale delibera del CIPE

260 interventi per un valore di 196 miliardi di euro, a moneta attuale. Quante di queste risorse si sono trasformate in cantieri aperti e avviati? La loro entità attuale - dati ufficiali del Ministero dell'economia e del Ministero delle infrastrutture - è un po' meno di 8 miliardi di euro: cento del programma iniziale dopo cinque anni. Ma più dei numeri, sul quale si sono esercitati, invece, dicendo cifre del tutto prive di fondamento, i senatori a cui ho fatto riferimento, contano le opere, i cantieri aperti, quelli semiaperti, quelli inaugurati, ma non aperti, quelli inaugurati e reinaugurati, ma non aperti, quelli appena progettati e quelli solo approvati in linea tecnica.

Cominciamo dal Mezzogiorno. Il blocco della autostrade siciliane promesse: c'è solo un piccolo tratto sulla Catania-Siracusa, peraltro, come ricorderete, immediatamente fermato dal crollo del viadotto di accesso all'autostrada, che è anche costato diverse vite. Nulla sulla Ragusa-Catania, neppure il progetto. Niente sulla ferrovia Messina-Palermo, ancora ferma nella galleria sotto i Nebrodi. La statale ionica in Calabria, che dovrebbe congiungere Reggio-Calabria con Taranto: nessun cantiere aperto, è solo avviata la progettazione La Salerno-Reggio-Calabria: cantieri aperti per il 3 per cento dei lavori preventivati; ferma al secondo lotto tra Atena e Lagonegro, come sanno tutti coloro che si recano in quella zona

dell'Irpinia: promessa e non ancora nemmeno messa in progettazione preliminare. La ferrovia di alta velocità Napoli-Bari: esiste solo la progettazione preliminare e nessun cantiere aperto. Il grande Il grande raccordo anulare di Roma (basta percorrerlo in questo periodo per verificare che taboga sia diventato dopo essere stato inaugurato addirittura per due volte dall'ex primo ministro Berlusconi). L'autostrada tirrenica tra dire, Civitavecchia e Genova, cioè l'autostrada che doveva essere realizzata e che per intervento prima dell'ex ministro Lunardi e poi dell'ex ministro Storace ha subito modificazioni tali che oggi non ha più nemmeno il progetto preliminare.

strada più cara del mondo, progettata dall'ingegner Lunardi: costa per metro lineare più del *tunnel* sotto La Manica), non ancora terminata. L'alta velocità Roma-Napoli, che è solo un'infrastruttura di campagna e non contiene né il nodo di Napoli, né quello di Roma. La Grosseto-Siena-Arezzo-Fano,

la ferrovia sul Brennero; i nodi di Firenze e Bologna; la ferrovia di alta velocità tra Milano e Venezia, ferma a Treviglio da tre anni; il terzo valico Genova-Milano, su cui si è esercitato il senatore Grillo e per il quale c'è soltanto un progetto preliminare che prevede un *project financing* che ne coprirebbe solo il 10 per cento la BreBeMi, che nonè mai iniziata; la tangenziale est di Milano, per la quale abbiamo dovuto trovare noi i soldi in questa finanziaria; la pedemontana lombarda; la gronda di Genova che non c'è; la Verona-Venezia-Padova. Mi voglio fermare queste sono le opere promesse e per le quali non c'è niente. L'ISPA, di cui tanto si è parlato ieri,

Non parlo di quanto è accaduto nei sedimi aeroportuali, dove tutte le promesse con le quali erano maturati, le trasformazioni delle concessioni concessioni da sei anni a quarantacinque anni, con una lievitazione enorme dei valori, non hanno prodotto nessuna pista in più e nessuna «testa di aeroporto» in più. Ora queste aspettative inevase, che avete sollecitato per cinque anni senza realizzarle, si scaricano sul disegno di legge finanziaria in esame e su questo Governo; voi vorreste speculare su questo e pretendere che noi facciamo in sei mesi quello che voi non avete saputo fare in cinque anni. Questa è una pretesa veramente assurda. tutti insieme riflettere sul sostanziale fallimento che ha registrato la finanza di progetto. Se si vanno a vedere i quantitativi di risorse private che in questi anni sono stati immessi nel sistema di finanziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie, si vede che la loro rilevanza è pressoché trascurabile. Tutte le opere sulle quali doveva intervenire la finanza di progetto sono ferme; la più significativa tra queste, l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano, doveva diventare un'autostrada interamente finanziata con risorse private, ma non ha nemmeno visto l'avvio del progetto definitivo. Senza il coinvolgimento di queste risorse del sistema privato, difficilmente si avranno risultati. Occorrerebbe procedere a una modifica delle norme, ma non se ne vede una traccia visibile nella legge finanziaria. Probabilmente su questo ci saremmo dovuti esercitare, non su ragionamenti di tipo propagandistico, che non fanno vedere qual è la verità delle cose e sicuramente ritardano la soluzione dei problemi infrastrutturali.

il tono, ma anche la genericità e il taglio un po' propagandistico dell'opposizione su questa finanziaria. Credo che, piuttosto che ragionare attorno a queste opposizioni,

il Presidente della Commissione bilancio del Senato. Non c'è dubbio: siamo in presenza di un'assoluta incongruenza tra gli strumenti di governo dell'economia e l'organizzazione della struttura democratica del nostro Paese. Non c'è soltanto il problema dello slittamento dalla legge di bilancio alla legge finanziaria, con la prima che si assottiglia e la seconda che diventa una sorta di *omnibus*; anche un problema vero, che riguarda il rapporto tra il Governo e il Parlamento, tra il ruolo dell'Esecutivo e il ruolo del Parlamento.

disgraziatamente e sciaguratamente si apprestava a fare il disegno di riforma bocciato giustamente dagli italiani con il *referendum*. Tale problema riguarda il rapporto tra lo Stato centrale, le Regioni e le autonomie.

finanziaria figli di questo coacervo di organizzazioni istituzionali, che non hanno una fisionomia e una responsabilità definita. Per cui le domande finiscono con lo scaricarsi tutte nell'occasione della predisposizione del bilancio e della legge finanziaria

Lo Stato sulla materia della sanità può intervenire, e interviene, a tagliare o a imporre il *ticket*, ma non è nelle condizioni di intervenire sull'organizzazione della struttura sanitaria e non è in grado neppure di richiamare le Regioni a una modalità di organizzazione della struttura che sia compatibile con i costi di un servizio che deve avere una dimensione sociale. Sotto questo profilo (la dico così), non è accettabile per nessun cittadino pagare un *ticket* quando si sa che un *manager* della sanità - considerato una specie di plenipotenziario e onnisciente, anche se molto spesso sappiamo che non lo è - guadagna 250.000 euro l'anno,

dalla gente in carne e ossa, da quella che vive i problemi quotidiani e non soltanto da quella parte della popolazione che difende in qualche modo una condizione acquisita, che può anche essere ritenuta di privilegio o frutto di un certo lassismo con cui si è considerato il dovere del contribuente nei confronti dello Stato, anzi, si è rappresentato lo Stato come una sorta di vampiro da cui

collettività la risposta a determinati problemi (dalla salute all'istruzione, dalla casa al lavoro).

l'assemblea della FIAT, i pronunciamenti e le preoccupazioni dei lavoratori rispetto a programmi prospettati, in realtà, più come minacce.

che vanno da quelli che conosco più direttamente, come la privatizzazione della Centrale del latte di Roma, fino a quelli più consistenti.

come le Ferrovie dello Stato, dove l'azionista unico sostanzialmente è lo Stato, non vi è bisogno di fare un presidente: basta un amministratore, ammesso che sia capace di farlo.

Il gradimento sulla potenzialità della nuova coalizione di Governo è fortemente ridimensionato dalle ampie critiche di una estesa parte della società circa le dinamiche politico-economiche attinenti alle aspettative e di consumo per le famiglie e di riforme strutturali per la competitività del Paese. Ciò appare chiaro anche dalla manovra finanziaria che contiene interventi disomogenei e discutibili, perfino sul piano costituzionale; non contempla alcuna prospettiva strategica ed è incentrata per due terzi sull'approvvigionamento di risorse attraverso l'inviso meccanismo della tassazione, senza beneficio per il contenimento della spesa pubblica; mentre si evidenzia una cospicua provvista da distribuire con la antica e dannosa tecnica dei privilegi ai più fedeli. E', quello delle tasse, un problema di cui chiunque abbia avuto a che fare con un testo di diritto tributario o di scienza delle finanze conosce lo svolgimento applicativo, i cui risultati apprezzabili fanno riferimento all'affidamento dello sviluppo dei tributi ordinari e non alla istituzione di imposte straordinarie, anche se, una volta applicate, promettono di restituirle, come vanno giustificandosi alcuni responsabili della politica di questo Governo. regola economica, invece, che all'aumento delle entrate debbano contribuire le imposte dirette e per avere un esito positivo, oltre che una buona sorveglianza ed una maggiore severità negli accertamenti, è necessaria anche una riduzione delle aliquote allo scopo di contenere l'incentivo all'evasione. Scelta messa in atto con successo altrove, e da noi la riduzione delle tasse operata dal Governo Berlusconi, pur in anni di travagli internazionali, ha generato, con la finanziaria 2004 e 2005, un gettito delle entrate così imprevisto da abbassare lo sforamento dei parametri di Uno dei nostri padri costituenti nel 1948 acclarava il principio per cui l'imposta è il fondamento primo sul quale si regge l'organizzazione dello Stato moderno, libero e democratico. E proprio al Senato, il 25 Luglio del 1950, l'onorevole Vanoni dichiarava: «Si deve essere molto perplessi ad insistere in un aumento delle entrate se esso deve essere destinato a spese di puro consumo». Sono insegnamenti ed esperienze che il Governo Prodi ha dimenticato, facendosi promotore di un aggravio della pressione fiscale che non ha precedenti in nessun Paese democratico, con soluzioni banali, sebbene vessatorie, come tutte quelle che mettono in atto coloro che scelgono il dirigismo, figlio di visioni totalitarie che hanno generato solo pauperismo e minimalismo nei confronti di quella platea sociale che, sebbene già nota al fisco, diviene oggetto di un odioso spionaggio fiscale con la massima trasparenza e nella legalità della legge che lo impone. Ci troviamo di fronte a norme inique che pur avrebbero una loro giustificazione se avessero come elemento teleologico il risanamento del Paese, con una strategia di investimenti in opere strutturali come avviate nel precedente Governo Berlusconi, egregio senatore Brutti Paolo. Purtroppo, non appare strategia alcuna, se non la solita indicazione generica di ridurre quel *deficit* pubblico che, da quando agli inizi degli anni Ottanta divenne trasparente, nessuno è più riuscito a dimensionare su base europea. Esiste, invece, una preoccupazione in quanto il debito pubblico è composto per buona parte da debito verso investitori esteri e questo Governo, nel modo più incauto, ha innalzato il prelievo fiscale sulle operazioni finanziare al 20 per cento, provocando il declassamento del nostro *rating*, senza porre attenzione al fenomeno della bassa tassazione applicata nei Paesi «ex cortina di ferro» che sono entrati a far parte di recente dell'Unione Europea e che rappresentano un fertile terreno di investimenti. Nei rapporti, poi, con i cittadini si constata l'ennesimo *vulnus -* lo abbiamo detto molte volte in Aula - ai dettami dello Statuto del contribuente, in quanto alcune norme tributarie, presenti anche nel collegato alla finanziaria, producono effetti retroattivi. Aspetto delicato, se si considera che la disattesa governativa non è solo formale o da considerarsi come un modo arrogante per fare cassa, fermo restando, ed è bene sottolinearlo, che a questa becera prassi non si prestano né la Guardia di finanza, né gli uffici finanziari ispettivi; ma è un metodo, quello del Governo, per pasticciare le decisioni delle aziende in ordine ai bilanci approvati precedentemente alle norme attuali. Il Presidente della Commissione bilancio ha mostrato una apprezzabile onestà intellettuale; ma non si può nascondere un evidente imbarazzo quando la maggioranza deve per forza approvare il provvedimento del Governo che contesta sé stesso presentando ben 160 emendamenti, con il supporto di altri 49 del relatore e centinaia della stessa maggioranza. Il perché di questo comportamento fa riflettere su un elemento inquietante nella gestione della finanza pubblica, rappresentato dall'occultamento di notizie circa l'andamento dell'economia con il fine di inculcare nell'opinione pubblica una presunta situazione disastrosa dei conti dello Stato. Ma occultare in politica è una scelta praticata anche quando governanti accorti costruirono la prima Repubblica, utilizzando la burocrazia e gli strumenti economico-finanziari creati durante il Ventennio e dei quali era impossibile discutere, soprattutto nella scuola dove si formava la nuova generazione, al punto che ancora nel 1970 quei giovani si domandavano perché sui registri a rigoroso rendiconto del Ministero delle finanze insistesse il logo della monarchia unito al simbolo del fascio. Si nascondeva alla massa che INAM, IRI, IMI, ENI, INAIL e tutta la burocrazia che fece da sostrato ai cinquanta Governi della durata media di non più di un anno venivano dal regime abbattuto dal sacrifìcio del popolo italiano. E l'attuale Governo è figlio di quella metodologia che riporta indietro il Paese di decenni tramite la responsabilità del Ministro delle finanze che non è un politico, e ciò in parte lo giustifica su certe sue improvvide dichiarazioni; il fatto poi che sia un professore acclara il detto popolare su coloro che predicano bene e razzolano male. Infatti, la nota presentata dal Governo in Commissione bilancio dimostra che le maggiori entrate incassate dall'erario a fine novembre 2006 superano di 34 miliardi le stime contenute nei dati di finanza pubblica. Il che significa che l'eredità lasciata dal Governo Berlusconi, riguardo al *deficit*, è del 2,1 per cento del 1992. Ne deriva che la finanziaria al nostro esame è concentrata su inasprimenti fiscali per soddisfare la richiesta di spesa pubblica dell'attuale maggioranza e realizzata con un falso bilancio, in quanto basata con saldi garantiti dal celato gettito fiscale aggiuntivo e non dagli interventi di finanza pubblica. E' una situazione preoccupante che rivela un accanimento fiscale dovuto all'ossequio che il Presidente del Consiglio deve alle liste radicali della sua coalizione; quell'intellighenzia che insiste sull'esperienza che ha fallito nei Paesi costretti al socialismo reale. L'evasione è la tabe di ogni società organizzata fatta di grandi numeri

La seduta è tolta